3 marzo 2009 Seguito della discussione del disegno di legge: (1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati)

L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonche´ ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

In data 25 febbraio 2009, il dottor Francesco Amirante ha inviato la seguente lettera: «Illustre Presidente, ho l’onore di comunicarle, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 87 del 1953,

come quello di Presidente della Corte costituzionale. Sospendo la seduta in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.

Questa mattina riprenderanno le votazioni sugli articoli e gli emendamenti al disegno di legge collegato in materia di semplificazione del processo civile. Come preannunziato alla Conferenza dei Capigruppo, l’articolo 26-quater, concernente delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, e stato nuovamente trasmesso alla 5ª Commissione permanente per il parere al Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. La Commissione bilancio dovrapronunziarsi entro l’inizio della seduta pomeridiana di oggi. Collega, la sua voce si sente fino a qui; la prego, sto leggendo il calendario. Nel corso di questa settimana, a conclusione del predetto disegno di legge collegato, si esaminerail decreto-legge in materia di produzione lattiera,

Per quanto riguarda il disegno di legge sul testamento biologico, per il quale il calendario corrente prevedeva l’avvio della discussione giovedı 5 marzo, alle ore 11, estato ritenuto opportuno ampliare i tempi di esame presso la Commissione competente. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo definito dalla Commissione o, in alternativa, al testo base del relatore e stato differito alle ore 12 di venerdı13 marzo,

Le votazioni degli emendamenti inizieranno a partire dalla seduta antimeridiana di martedı24 marzo. La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedı 10 marzo, con inizio alle ore 18, saradiscussa la relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica sui dati sensibili. Nel dibattito, che si concludera – secondo i precedenti – senza votazione di strumenti, potranno intervenire, dopo la relazione introduttiva, un oratore per Gruppo ed il Governo. Nel corso di tale settimana si passerapoi all’esame del disegno di legge comunitaria 2008 e dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali definiti dalla Commissione Nella prossima Conferenza dei Capigruppo, da convocarsi all’inizio della prossima settimana, sara presa in considerazione la mozione preannunziata dal Gruppo del Partito Democratico, ai fini di un dibattito sulla crisi occupazionale.

come preannunciato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, alla luce delle osservazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro e dai senatori Morando e Legnini, ha trasmesso nuovamente alla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, l’articolo 26-quater in materia di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Avverto che sono da ritenersi improponibili per estraneitaalla materia gli emendamenti aventi ad oggetto il coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, norme interpretative della disciplina concernente l’attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali, l’istituzione di organismi di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l’istituzione di organismi di vigilanza sulle risorse idriche.

darle atto della decisione che lei ci ha appena comunicato, che corrisponde ai rilievi che noi avevamo formulato in punto di applicazione del nostro Regolamento,

costituisce un contributo al corretto svolgimento dei nostri lavori, cosıcome avvenne sulla materia, del tutto analoga, dell’ammissibilita degli emendamenti ai decreti-legge, con la decisione che lei ebbe a comunicare nella seduta

Informo l’Assemblea che sono presenti gli studenti della scuola media statale «Don Salvatore Vitale» di Giugliano, in provincia di Napoli.

Abbiamo appreso ora che il Governo sta presentando un decreto-legge sui precari, che annullerebbe le norme presenti nel suddetto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti: «8-bis. All’articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma e` sostituito dal seguente:

Il giudice ha sempre facolta di disporre la rinnovazione delle indagini e, per inosservanza dei termini di cui all’articolo 195 o per altri gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. Il giudice dispone, con decreto che costituisce titolo esecutivo, la restituzione dei compensi riscossi dal consulente sostituito”».

alle controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento. Il comma 1-bis stabiliva che la materia fosse trat dal giudice di pace, non applicando chiaramente il rito del lavoro, ma nulla diceva per quello che riguardava la fase dell’appello.

proposte volte ad aumentare le competenze dei giudici di pace per quanto riguarda le cause civili di sinistri stradali. 3 marzo 2009 sente che anni fa, quando finalmente si riuscıa fare un inventario delle cause civili, si stabilı

di dedicare maggior tempo alle cause civili, di eliminare un arretrato immenso e, soprattutto, di ridurre i tempi di definizione dei processi, che lo stesso Ministro ha avuto occasione di

e per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino al limite di 20.000 euro. Inoltre, e stata aumentata la competenza per valore in tutte le

tribunale ordinario ed il giudice di pace. Pertanto, la misura indicata ci sembra un giusto bilanciamento di lavoro tra le due giurisdizioni.

come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 - stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari si applicano fino a quando non sara` attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009; il disegno di legge AS n. 1082/A amplia la competenza dei giudici di pace nelle controversie in materia civile;

per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del giudice di pace; si rende improcrastinabile una riforma organica dell’intera magistratura onoraria al fine di razionalizzarne l’impiego nell’organizzazione del servizio giustizia impegna il Governo a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, valutando l’opportunita` di prorogare i giudici di pace in servizio a tale data qualora non fosse ancora concluso l’iter parlamentare di approvazione della riforma».

introdurre per cercare di definire le controversie alla prima udienza, dando al giudice la possibilita di ordinare la comparizione delle parti e di tentare la conciliazione.

ritiro, signor Presidente.

le chiedo il permesso di illustrare, anche se molto rapidamente, il significato di tale proposta, che era gia` prevista all’articolo 26, in forme analoghe e a firma di altri sottoscrittori, senatori della maggioranza e dell’opposizione.

l’emendamento 28.700 del Governo, che riguarda questo argomento, mi pare che proponga di sostituire le parole «raccolta dal difensore» con le seguenti:

consegnare la testimonianza scritta al difensore. Pertanto, abbiamo aggiunto «esaminate le risposte o le dichiarazioni» nell’ipotesi in cui fosse consegnata direttamente la testimonianza al difensore. Si tratta soltanto una specificazione tecnica. senatore Benedetti Valentini per

intervengo solo ad adiuvandum. Voglio far presente ai colleghi e al Governo che la formula «ricevere» eutilizzata dal codice civile e dalla legge sul notariato per qualificare l’atto pubblico.

Presidente, mi edispiaciuto che il senatore Benedetti Valentini abbia rinunciato ai suoi emendamenti, che proponevano di abolire

era davanti alla pretura chi affittava la giacca per il testimone falso. Mi domando cosa succede quando si delega

la giuria viene formata proprio per raccogliere la prova; bisogna che il teste vada davanti alla giuria e faccia una dichiarazione, a meno che non si riconoscano determinati fatti.

Presidente, vorrei chiarire all’Aula, dopo l’intervento del collega D’Ambrosio, che questa prova puoessere disposta

prova. Non vi e alcuna rinuncia immediata alla giurisdizione o al controllo sulle dichiarazioni testimoniali.

Dichiaro aperta la votazione.

Presidente, l’emendamento 28.40 nasce dal fatto che io propendo sempre per la sostanza piuche per la procedura.

siccome nel nostro sistema processuale resta in piedi la norma secondo la quale il giudice anche d’appello, sol che lo ritenga indispensabile ai fini della decisione e allorche´ magari vi sia la prova

Non epossibile immaginare che un ricorso per Cassazione venga dichiarato inammissibile inaudita altera parte, senza nemmeno avviare una procedura di verifica nel contraddittorio dei soggetti processuali.

la sezione che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente dei ricorsi inammissibili. Il numero di di ricorsi che vengono dichiarati inammissibili enotevole, ma se ne discute, signora Presidente; e prevista la possibilitadi intervento da parte dei soggetti L’ipotesi che si vuole introdurre con l’emendamento 29.4 e volta ad evitare che una sezione di tribunale diventi una sorta di commissione che svolga delle valutazioni senza ascoltare il parere di alcuno, sulla base di considerazioni che non potranno mai essere censurate perche´ poi naturalmente non esiste un’istanza ulteriore. Credo che il rispetto del contraddittorio,

con questo emendamento si era aperto in Commissione il confronto, amplissimo, sul problema dell’ammissibilitadel ricorso per Cassazione. E[ ]stato svolto un cospicuo ed approfondito lavoro nella sede delle Commissioni stesse e ritengo giusto attenermi al non facile risultato del dibattito e del comune lavoro in Commissione. Sottolineo, in particolare, che con la soppressione

Presidente, accolgo l’invito al ritiro, pero` non posso esimermi dal fare una considerazione amara: talvolta si ha l’impressione che l’agenda dei nostri lavori sia scandita da esigenze della Cassazione.

(PD). Chiediamo la verifica del numero legale.